la mozione ricostruisce molto pacatamente una vicenda della quale si è parlato a lungo in queste ultime settimane.

il Supremo tribunale federale (STF) ha dichiarato nullo il provvedimento di rifugio, concesso l'estradizione richiesta dall'Italia e autorizzato il Presidente brasiliano a consegnare Cesare Battisti al nostro Paese, in conformità al vigente Trattato bilaterale in materia di collaborazione estradizionale, una pagina di onore di quel Trattato. La situazione poi, proprio nelle ultime settimane, ha avuto un improvviso rovesciamento: l'Avvocatura generale dello Stato brasiliana ha reso pubblico un proprio parere, formulato all'ex Capo dello Stato brasiliano, che, in forza di un articolo del Trattato bilaterale,

citato - viene riportato nella mozione. L'Avvocatura generale del Brasile ha sostenuto che l'estradizione non viene concessa «se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua». Come voi capite, pur trattandosi di un parere, non mancano implicazioni che offendono la storia, la realtà, la natura e le procedure L'Italia nei confronti di Battisti ha da far valere esigenze di giustizia non esigenze di vendetta, che sono estranee al nostro ordinamento. abbia molto ferito e intaccato nell'opinione di importanti giuristi la credibilità di quel Trattato. L'Italia però - l'opinione pubblica, almeno - non si rassegna a che sia così. Pertanto, attraverso questa mozione, condivisa, auspichiamo che il nostro Governo possa riprendere la trama su tutte le strade del versante giurisdizionale lasciate aperte dal Supremo tribunale federale, come previsto da un punto della mozione sul quale sarà interessante ascoltare le valutazioni del rappresentante del Governo, di adire eventualmente la Corte internazionale di giustizia, affinché il rifiuto opposto dall'ex Presidente brasiliano alla concessione dell'estradizione venga rimosso. Ripeto, il senso della mozione è di impegnare il Governo ad assicurare Cesare Battisti alla giustizia italiana, proprio in nome del procedimento previsto dal Trattato bilaterale. Di qui la nostra fermissima intenzione di dare voce a quei sentimenti e a quegli argomenti dell'opinione pubblica secondo quel Trattato e, soprattutto, le buone relazioni con il Brasile possono ancora recuperarsi. Proprio per tali ragioni, con lo spirito non di una minaccia minaccia ma di percorrere tutte le prospettive che si aprono sul versante della giurisdizione, la mozione formula anche l'ipotesi di adire la Corte internazionale di giustizia. Questo è il

perché stiamo trattando di una vicenda che oggettivamente - possiamo dirlo con serenità - sta offendendo il nostro Paese, Paese, le tante vittime del terrorismo, i loro familiari e tutti gli italiani. Il Presidente brasiliano, come tutti sappiamo, sappiamo, nonostante le numerosissime sollecitazioni che gli sono arrivate a livello internazionale, ha scelto di negare l'estradizione di Cesare Battisti. relatore, sulla decisione del Presidente del Brasile molta influenza ha esercitato l'Avvocatura generale, con un parere in cui sostanzialmente si raccomandava di negare l'estradizione di Cesare Battisti.

l'Avvocatura ha argomentato il suo parere al Presidente brasiliano sostenendo che, se Battisti ritornasse in Italia, potrebbe trovarsi in una grave situazione.

Battisti è innocente, che non ha niente a che vedere con gli omicidi per i quali - lo ricordiamo - è stato condannato con sentenza passata

addirittura arrivando ad affermare che l'accusa di omicidio nei confronti di Battisti fu mossa da persone di dubbia attendibilità. È chiaro che ci troviamo di fronte a una decisione inaccettabile, a una lettura della storia inaccettabile. E, quindi, è bene che oggi il Parlamento italiano, in particolare

in questo caso, come usa dire, *bipartisan*, che veda una convergenza assoluta di tutte le forze politiche, in cui si impegna il Governo ad assumere una serie di iniziative:

del rispetto dei sentimenti, come ho già detto all'inizio del mio intervento, delle vittime, dei loro familiari e di tutti gli italiani. Come sappiamo, cari colleghi, in alcune Assemblee legislative regionali e enti locali si stanno

europei dell'Italia dei Valori, è stata presentata un'interrogazione alla Commissione competente e una risoluzione che andrà in discussione proprio questa settimana, anche in considerazione del fatto che il Parlamento europeo si è espresso già su tale questione, il 5 febbraio 2010, ponendo in evidenza che la questione legata all'estradizione di Battisti ha una rilevanza a livello europeo, perché riguarda il riconoscimento dei sistemi di giustizia degli Stati membri da parte del Brasile.

Sud-MRE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la mozione presentata intendiamo prendere posizione e condannare fermamente la decisione dell'allora presidente della Repubblica Federativa del Brasile, Lula, di negare l'estradizione di Cesare Battisti, pluricondannato per omicidio e reati di terrorismo in Italia. Tale decisione desta meraviglia alla luce delle importanti relazioni di amicizia tra Italia e Brasile e desta altrettanta meraviglia la motivazione con la quale è stata presa. Infatti, gli argomenti addotti sono contrari al trattato di estradizione vigente tra i due Paesi, sembrano superficiali e infondati nel merito. Cesare Battisti è stato definito «agitatore politico che operò negli anni diffìcili della storia italiana, e che, sebbene condannato per crimini di matrice comune, potrebbe subire conseguenze negative dalla sua estradizione». È stato affermato dagli organi istituzionali del Brasile che, a seguito dell'estradizione, «ci sono ponderate ragioni per ipotizzare che il detenuto potrebbe soffrire forme di aggravamento della sua situazione». Voglio brevemente in questa sede ripercorre la storia personale e giudiziaria del terrorista Cesare Battisti negli anni di piombo, affinché non si dimentichi o non si sottovaluti il personaggio in questione. Nel fare ciò vorrei anche rivolgere un omaggio alla memoria di quanti ne sono stati vittime e un pensiero anche alle loro famiglie. Cesare Battisti, inizia la sua carriera criminale nel 1971. Venne per la prima volta arrestato nel 1972 per una rapina compiuta a Frascati. Nel 1974 venne nuovamente tratto in arresto per una rapina e sequestro di persona. Nel 1977 di nuovo arrestato, sempre per rapina, e in carcere entrò in contatto con i Proletari armati per il comunismo In Italia Cesare Battisti è stato condannato come responsabile di quattro omicidi, reati evidentemente di matrice comune: tre come concorrente nell'esecuzione, uno come coideatore ed eseguito da altri.

Milano. Nel 1979, Battisti venne arrestato nell'ambito di un'operazione antiterrorismo di vaste proporzioni e detenuto nel carcere di Frosinone. Il 4 ottobre 1981 Battisti riuscì ad evadere e a fuggire a Parigi, per poi trasferirsi in Messico. Durante la sua latitanza messicana, i giudici italiani lo condannarono in contumacia all'ergastolo perché giudicato responsabile dei quattro omicidi e di varie rapine. Tornato a Parigi, viene arrestato a seguito di una prima richiesta di estradizione del Governo italiano, ma nell'aprile dello stesso anno è dichiarato non estradabile. Il 10 febbraio 2004 venne nuovamente arrestato a Parigi e la magistratura italiana chiese, ancora una volta, la sua estradizione, che venne concessa dalle autorità francesi il 30 giugno 2004. A seguito del provvedimento francese, Battisti, che nel frattempo godeva della libertà vigilata, si rese latitante, lasciando la Francia e facendo perdere le sue tracce. Venne poi arrestato a Copacabana, in Brasile, il 18 marzo 2007. Il 13 gennaio 2009, il Brasile decise di accordargli lo *status* di rifugiato politico, motivando la decisione su quello che viene definito «il fondato timore di persecuzione del Battisti per le sue idee politiche». tesi tutt'oggi, come già detto, è a fondamento della decisione che ha portato l'ex presidente Lula, nell'ultimo giorno del suo incarico, il 31 dicembre 2010, ad esprimersi contro l'estradizione di Battisti. Su questo caso si sta impegnando anche il Parlamento europeo. È notizia della scorsa settimana (13 gennaio) che giovedì prossimo (20 gennaio), l'Aula di Strasburgo discuterà e voterà una risoluzione *bipartisan*, presentata dai due Vice Presidenti italiani del Parlamento europeo e sottoscritta da tutti i Gruppi politici per chiederne l'estradizione. Oggi la politica deve far sentire il suo peso e la sua determinazione affinché il timore, espresso anche dal presidente Napolitano, che si disperda la memoria dell'attacco terroristico alla Repubblica, non divenga reale. Il nostro Presidente della Repubblica ha anche detto: «È mancato qualcosa alla nostra cultura e alla nostra politica per trasmettere e far capire davvero il senso di ciò che accadde in quegli anni tragici del terrorismo». Alla luce di quanto accaduto, la politica non può mostrarsi debole e ha il dovere di ricordare e di dare valore alla forza straordinaria che è servita per battere quell'infausta esperienza. Signor Presidente, è per questi motivi che oggi, quindi, chiediamo con fermezza al Governo che si impegni a promuovere ogni opportuna iniziativa presso il Tribunale supremo federale del Brasile, presso la Commissione di conciliazione istituita ai sensi del vigente accordo bilaterale tra Italia e Brasile e presso la Corte internazionale di giustizia ONU dell'Aja e in ogni altra sede istituzionale o giurisdizionale competente, affinché, ricercando ogni soluzione condivisa con la Repubblica Federativa del Brasile, si pervenga all'estradizione nei tempi più celeri possibili di Cesare Battisti in Italia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il Presidente della Repubblica nei giorni scorsi ha detto che sul caso Battisti forse, come Paese, non ci siamo fatti capire a sufficienza: non siamo riusciti a spiegare ad amici vicini e lontani cosa è stata quella che il collega Zavoli, in una celebre trasmissione televisiva, definì "la notte della Repubblica", la lunga stagione del terrorismo che ha insanguinato il nostro Paese.

non c'è un regime che si difende, ma un Paese che si considera offeso da una decisione che non capisce. Il Brasile è un Paese amico, è un Paese amico, impregnato di presenza e di cultura italiana, ed è anche un Paese con il quale abbiamo interessi commerciali importanti per lo sviluppo di entrambi i nostri i nostri sistemi economici. È un Paese amico e, in particolare noi democratici italiani, abbiamo simpatizzato e solidarizzato a lungo, per anni, con il presidente Lula per la sua dura e coraggiosa lotta, prima sindacale - è stato il *leader* di un grande movimento sindacale che ha cambiato le relazioni industriali in Brasile - e poi politica, per la democrazia e la giustizia sociale in quel Paese. in quel Paese. È proprio per questo che siamo rimasti senza fiato di fronte alla decisione di negare l'estradizione di Cesare Battisti. una decisione che consideriamo sbagliata sul terreno giudiziario, come si spiega con efficacia nella mozione, ma soprattutto ingiusta sul piano politico e morale, perché frutto di un abbaglio storico.

Battisti non è stato condannato da un tribunale speciale, ma attraverso sette processi che hanno coinvolto 24 magistrati italiani. La giustizia italiana è certamente imperfetta e ha molti limiti. Siamo noi continuamente a denunciarlo in queste Aule: la durata dei processi, un eccesso di ricorso alla carcerazione preventiva. Ma certamente, tra questi difetti, non ha quello di mancare di garanzie per l'imputato nel processo: semmai, eccediamo nel senso contrario. E la presidente Rousseff - ha detto Tarso Genro - «si è battuta con coraggio contro un potere tirannico, il potere di una dittatura militare, per il ritorno delle libertà democratiche». Ecco l'abbaglio storico: Battisti ha ucciso persone innocenti per rovesciare la democrazia in Italia. Ha fatto quindi esattamente il contrario. Si è battuto uccidendo persone innocenti per rovesciare le libertà democratiche, quelle libertà democratiche e quella democrazia che il popolo italiano aveva riconquistato con l'antifascismo e con la Resistenza, cioè al prezzo di dure lotte. L'Italia ha difeso la sua democrazia con lo Stato di diritto e dentro lo Stato di diritto, senza leggi o tribunali speciali, senza mai violare i diritti costituzionali e senza mai violare i diritti umani fondamentali. Questa è una pagina di cui noi andiamo orgogliosi. Noi siamo un Paese che spesso è molto critico su se stesso, e questa tuttavia è stata una pagina sofferta ma dalla quale l'Italia è uscita maturata, più consapevole, proprio perché ha saputo difendere la democrazia con la democrazia e con la libertà. Battisti ha violato questi valori e questi principi perché ha combattuto la democrazia con la violenza, e non può esserci nessuna giustificazione per chi usa la violenza contro la democrazia. La democrazia è sempre un regime imperfetto, ma è perfettibile. Questo implica come la lotta politica in democrazia si possa e si debba svolgere solo attraverso

di cittadini che la nostra Costituzione difende. Questo noi vorremmo far capire, con amicizia, al popolo brasiliano e a chi avrà, nelle prossime settimane e nei il compito di decidere su una vicenda che noi non consideriamo conclusa, proprio perché crediamo nell'amicizia con il popolo ed il Governo brasiliano. finestra"). È presente in Aula una delegazione di studenti della Scuola media statale «Gesualdo Nosengo» di Arzano, in provincia di Napoli. A loro va il saluto dell'Assemblea.

Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio innanzitutto rinnovare al popolo brasiliano, al Governo federale e a quello dello Stato di Rio de Janeiro i sentimenti di cordoglio per le vittime della tremenda alluvione che ha colpito il Paese e trasmettere ancora una volta ai familiari la solidarietà degli italiani. In questi giorni il nostro ambasciatore a Brasilia ha già presentato al Governo federale un *memorandum*, indicando le forme della collaborazione italiana per contribuire a far fronte alle drammatiche situazioni determinatesi. È questa la solidarietà di un popolo amico che ha coscienza dei profondi legami umani, culturali e politici tra i due Paesi: vincoli consolidati dalle decine di milioni di brasiliani i cui antenati hanno lasciato la nostra terra e hanno concorso al grande progresso del Brasile moderno. A quel progresso hanno contribuito tante imprese italiane; a quel progresso potremo continuare a partecipare proprio attraverso gli strumenti di cooperazione strategica in atto tra i due Paesi. È proprio in nome di questi profondi legami tra Italia e Brasile che in questo momento e nella sede più alta della rappresentanza popolare, il Parlamento, dobbiamo esprimere al Governo brasiliano, e certamente da amici, la nostra profonda amarezza e, in modo netto e senza equivoci possibili, il nostro dissenso per la decisione di non estradare, in base alle norme di un Trattato bilaterale, un cittadino italiano colpevole di gravi reati di sangue e condannato dai tribunali italiani nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali. Vorrei quindi esprimere apprezzamento per questa opportuna e tempestiva iniziativa che il Parlamento, in entrambi i suoi rami, ha inteso assumere per lanciare un ulteriore e forte segnale a testimonianza dell'attenzione con cui tutto il nostro Paese segue il caso Battisti. con alto senso delle istituzioni, approverà tra poco con voto unanime una mozione che chiede, con toni pacati ma ferma e unanime determinazione, che la vicenda possa finalmente concludersi con l'estradizione del cittadino italiano. A questi fini, il Governo, forte dell'impulso dell'intero Parlamento e del consenso dei cittadini, si impegna ad operare, come da tempo sta facendo, perché tale risultato di giustizia e civiltà possa essere raggiunto. La decisione di non concedere l'estradizione a Battisti ha infatti scosso profondamente l'opinione pubblica italiana perché offende la memoria delle vittime degli atti criminali di Battisti e la sensibilità dei loro familiari. Essa contraddice i principi basilari del diritto e sembra quasi mettere in dubbio l'affidabilità del nostro sistema giudiziario, ponendo quindi in discussione quello dell'intera Unione europea. È una decisione, per questi motivi, condannata dal Governo, ma anche da tutte le forze politiche di questo Parlamento, senza alcuna distinzione. L'Italia, che rispetta naturalmente la sovranità del Brasile e ha piena fiducia nell'indipendenza della magistratura brasiliana, ritiene assolutamente non corrispondente al diritto il diniego dell'estradizione. Nei mesi scorsi, tramite contatti ai massimi livelli e una costante azione della nostra ambasciata a Brasilia, che ha in questo senso ricevuto costanti e puntuali istruzioni dal Ministro degli esteri, erano state illustrate le ragioni e le aspettative del nostro Paese. Il Capo dello Stato, fino alle ultime ore prima della decisione, e il Governo hanno sempre sottolineato di confidare nel rispetto della decisione del Tribunale supremo federale di concedere l'estradizione a Battisti. Da ultimo, il 21 dicembre, il Sottosegretario alla Presidenza, su impulso del Presidente del Consiglio, aveva nuovamente, e non senza una certa fermezza, rappresentato all'ambasciatore del Brasile le attese italiane. Abbiamo quindi accolto con grande disappunto e profonda delusione la decisione dell'ex Presidente brasiliano. Disappunto e delusione che sono stati espressi con chiarezza ai nostri interlocutori a Brasilia. Cogliamo e coglieremo tutte le occasioni per rappresentare alle autorità brasiliane l'aspettativa che il vigente Trattato bilaterale di estradizione sia correttamente interpretato e applicato, e che quindi Battisti venga estradato in Italia. Percorreremo tutte le possibili vie giudiziarie. Signor Presidente, onorevoli senatori, la decisione dell'ex Presidente va, del resto, in senso contrario rispetto al precedente verdetto del Tribunale supremo federale. La più alta istanza giudiziaria del Brasile aveva, come noto, dichiarato nullo il provvedimento di rifugio. Aveva concesso l'estradizione richiesta dall'Italia e autorizzato quindi il Presidente brasiliano a consegnare Cesare Battisti al nostro Paese, in conformità con il Trattato bilaterale, pur precisando che la pronuncia faceva salve le competenze del Presidente stesso. Tali sviluppi già avevano fornito un eloquente e autorevole conforto, da un punto di vista giuridico, alle tesi da noi sempre sostenute, con convinzione e tenacia, in tutte le fasi di questa purtroppo lunga vicenda. Tesi sulle quali poggia, tuttora intatta, la consapevolezza delle nostre ragioni. L'Italia - pur in un quadro di relazioni bilaterali che intende preservare - continuerà quindi a battersi in nome di un'esigenza fondamentale di giustizia. Lo farà su tutti i piani e con tutte le modalità offerte dagli strumenti giuridici, di natura interna ed internazionale. Lo farà per difendere e promuovere gli interessi più alti dello Stato e la piena applicazione dei principi della certezza del diritto che rendono necessaria la condanna e l'assoggettamento a pena di quanti si siano resi colpevoli di crimini odiosi. Non intendiamo mettere in discussione la tradizionale collaborazione con il Brasile, una cooperazione articolata e mutuamente vantaggiosa. Milioni di nostri connazionali, è bene ricordarlo, sono divenuti cittadini brasiliani. Al popolo brasiliano, lo voglio ripetere, ci uniscono vincoli radicati nella storia e con esso intendiamo continuare a costruire forme di cooperazione politica, economica e sociale in conformità con gli accordi che abbiamo stipulato. Quello che noi vogliamo, lo ribadisco, è contrastare, con la massima determinazione, una decisione che riteniamo ingiusta e infondata. La nostra linea s'ispira, dunque, a fermezza e misura allo stesso tempo. mi fa piacere constatare che questo è l'approccio che ho registrato in quest'Aula. Atteggiamenti che contribuissero ad esasperare il clima non servirebbero a conseguire l'obiettivo e potrebbero anzi rivelarsi controproducenti: rischiamo paradossalmente di essere strumentalizzati. È bene tenere presente che il parere dell'Avvocatura generale dello Stato brasiliana - che noi contestiamo e su cui il Presidente uscente si è basato - invoca, senza fondamento, proprio quel passaggio del Trattato bilaterale che esclude l'estradizione ove l'estradato possa subire atti persecutori o discriminatori o comunque la sua situazione rischi di essere aggravata. Vogliamo ricordare ai nostri amici brasiliani la storia italiana e sottolineare come anche il terrorismo è stato sconfitto proprio grazie alla reazione ferma della comunità nazionale, ma sempre nel pieno rispetto delle regole dello Stato di diritto. Fermezza e misura, appunto, sono state la nostra stella polare anche nei passaggi più delicati. E voglio sottolineare come, nel caso di Battisti, siamo in presenza di reati comuni. Già all'indomani dell'annuncio della decisione del presidente uscente Lula, il Governo italiano si è mosso prontamente. Tramite i suoi legali si è subito opposto alla richiesta di scarcerazione depositata dagli avvocati di Cesare Battisti. Il Tribunale supremo federale ci ha dato ragione e ha respinto, lo scorso 6 gennaio, l'istanza di liberazione, con una pronuncia che dà ulteriore conferma alle nostre tesi. Viene escluso che la giurisdizione dell'Alta corte brasiliana sia esaurita; viene ricordato che a suo tempo il Tribunale supremo federale aveva riconosciuto «l'assoluta assenza di prove di rischio di persecuzione politica» nei confronti di Battisti; si ribadisce che la discrezionalità della decisione presidenziale era subordinata al rispetto del Trattato bilaterale limitatamente alla consegna dell'estradando; viene negata la presenza di fatti nuovi che possano indurre a ritenere l'esistenza di «ragioni ponderate per supporre che la persona richiesta sarà soggetta ad atti di persecuzione e discriminazione» una volta estradata. L'impugnazione incidentale, subito accolta dal Tribunale supremo federale, prelude peraltro al vero e proprio ricorso che avanti a quella stessa Corte ci accingiamo a presentare. In vista del riesame del caso, il ricorso di diritto interno brasiliano per annullare il rifiuto dell'estradizione sarà avverso il parere dell'Avvocatura generale, che presta il fianco a più di un'obiezione, difettando di coerenza e profondità giuridica, e la decisione dell'ex Presidente, che si limita a recepire senza commenti o motivazioni il parere stesso. Esso verrà presentato, per motivi di opportunità, nell'imminenza della riapertura dei lavori del Tribunale supremo federale prevista a fine febbraio. Confidiamo nella solidità delle nostre argomentazioni, ma non vogliamo certo farci trovare impreparati, nemmeno di fronte alla più negativa delle prospettive. Nella malaugurata ipotesi che il ricorso di diritto interno brasiliano non avesse successo, sarà infatti possibile esperirne uno alla Corte internazionale di proprio perché la mancata estradizione di Cesare Battisti appare configurare una violazione del Trattato bilaterale italo-brasiliano del 1989 da parte del Brasile e la sua conseguente responsabilità sul piano internazionale. Inoltre, poiché Italia e Brasile sono vincolati dalla Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario del 1954, si potrebbero - come è stato ricordato in questa Aula - anche esperire i mezzi di soluzione delle controversie previsti da tale accordo per ottenere l'accertamento, da parte di un terzo imparziale, della sussistenza di una violazione. La Convenzione del 1954 stabilisce, infatti, che le «controversie di qualunque natura» sorte tra le parti e non risolte per via diplomatica possano essere sottoposte ad un procedimento di conciliazione. Il procedimento si conclude con una proposta da parte del conciliatore che le parti sono libere o meno di accettare. Se il tentativo fallisce, ciascuna delle due parti può adire unilateralmente la Corte internazionale di giustizia. Qualora, infine, la Corte dovesse ritenere la controversia non giuridica, le parti potranno convenire che essa venga risolta *ex aequo et bono* dalla stessa Corte. Vorrei, infine, sottolineare che di fronte all'ingiusto diniego dell'estradizione di Battisti l'Italia si è subito attivata anche sul fronte europeo. Come accennavo all'inizio del mio alla base della decisione dell'ex presidente Lula rappresentano, infatti, una inaccettabile sottovalutazione non solo dell'ordinamento italiano, ma anche dell'intero sistema comunitario di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. È per questo motivo che nel corso delle ultime settimane, a seguito di un provvedimento che appare essere in totale contraddizione con la natura stessa dell'Unione europea di comunità fondata sul rispetto del principio dello Stato di diritto e con gli elevatissimi livelli delle garanzie e delle tutele riconosciute dagli ordinamenti di tutti i Paesi membri, abbiamo provveduto a sensibilizzare anche i partner comunitari affinché sostengano le iniziative messe in campo dall'Italia volte ad ottenere l'estradizione di Cesare Battisti, nella consapevolezza che essa non può e non deve essere considerata una vicenda puramente bilaterale. Molto significativa è, in questo senso, una proposta di risoluzione presentata da vari Gruppi e già iscritta all'ordine del giorno della sessione plenaria di Strasburgo. La discussione dovrebbe avvenire questo giovedì. La risoluzione auspica che il nuovo ricorso italiano possa essere accolto dalle autorità competenti brasiliane e ricorda che il partenariato tra Unione europea e Brasile è fondato sul riconoscimento reciproco che entrambe le parti rispettano la legalità e i diritti fondamentali. Signor Presidente, il Governo è convinto che le pronunce del Parlamento nazionale ed europeo non potranno che rafforzare l'azione che l'Italia sta conducendo, al massimo livello e con la massima determinazione, per ottenere la giusta estradizione di Cesare Battisti contro il parere dell'Avvocato generale che motiva la decisione dell'ex Presidente. Noi ci auguriamo che anche da questa difficile prova esca rafforzata l'amicizia tra i due popoli e la cooperazione tra i due Governi.

Oggi parliamo purtroppo del cittadino italiano Cesare Battisti, che è stato condannato all'ergastolo, con sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano del 1988 e definitiva in Cassazione nel 1993, per omicidio plurimo, oltre che per i reati di banda armata, rapina e detenzione di armi.

24 giudici italiani ne hanno stabilito la colpevolezza. Sottrattosi alla giustizia italiana e rifugiatosi in Francia, Battisti è stato tratto in arresto l'11 febbraio 2004, in esecuzione di una richiesta di estradizione avanzata dalla giustizia italiana. Ma non appena Parigi si è pronunciata in senso favorevole all'estradizione, egli si è reso latitante. Nel 2006 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Battisti contro il provvedimento di estradizione concesso dalla Francia, stabilendo, tra l'altro, che i giudici italiani avevano perfettamente rispettato gli standard europei (quanto a diritto d'accesso e informazioni sul procedimento e diritti della difesa). Sulla base delle richieste sia italiana che francese, il 18 marzo 2007 Battisti è stato arrestato a Rio de Janeiro, e il 24 marzo dello stesso anno l'Italia ne ha richiesto l'estradizione.

concesso l'estradizione richiesta dall'Italia e autorizzato il Presidente della Repubblica brasiliana a consegnare Cesare Battisti al nostro Paese in conformità al vigente Trattato bilaterale in materia di collaborazione estradizionale, pur precisando che la pronuncia faceva salve le competenze del Presidente stesso; il Capo dello Stato, dalle cui dichiarazioni pubbliche e atti istituzionali il Paese si sente pienamente rappresentato, e il Governo italiano, nelle molteplici occasioni di contatto,

il 30 dicembre 2010, l'Avvocatura generale dello Stato brasiliana ha reso pubblico il proprio parere, approvato dal Vice Avvocato generale,

per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti»), si poneva in senso contrario alla concessione dell'estradizione di Battisti; il 31 dicembre l'ex Presidente della Repubblica brasiliana ha reso nota la propria decisione - conforme al parere dell'Avvocatura - che non accoglie la richiesta di estradizione dell'Italia nei confronti del connazionale; considerando poi in particolare che: la mancata estradizione di Cesare Battisti configura, nell'opinione di autorevoli giuristi, una violazione del predetto Trattato bilaterale di estradizione del 1989 da parte del Brasile, ciò che implicherebbe la responsabilità del Brasile sul piano internazionale per aver disatteso le disposizioni dell'accordo stesso; la decisione brasiliana di addurre come motivazione l'art. 3, lettera *f)*, del Trattato bilaterale di estradizione rende tale diniego profondamente ingiusto sul piano dei principi e infondato sul piano legale; il Presidente del Supremo tribunale federale del Brasile con decisione del 6 gennaio 2011 ha negato la scarcerazione di Battisti e inviato gli atti al giudice relatore per un ulteriore esame del caso in sede plenaria; il caso Battisti, infine, non sembra limitarsi ad una semplice questione bilaterale tra Italia e Brasile, in quanto, essendo che il sistema giudiziario dell'Italia sia in grado di offrire adeguate garanzie al condannato, il diniego dell'estradizione mette in discussione il rispetto dei principi stessi di civiltà giuridica da parte di tutta l'Unione europea, quale omogenea comunità di valori e spazio di libertà e giustizia, essendone l'Italia un Paese membro, impegna il Governo: a percorrere tutte le strade sul versante giudiziario offerte dal Supremo tribunale federale, non lasciandone intentata alcuna, fino ad adire, eventualmente, la Corte internazionale di giustizia e ogni altra sede istituzionale o giurisdizionale competente affinché il rifiuto opposto dall'ex Presidente brasiliano alla concessione dell'estradizione venga rimosso e Cesare Battisti possa essere assicurato alla giustizia italiana, a completamento del procedimento estradizionale, come previsto dal Trattato bilaterale e affinché sia ricercata ogni soluzione condivisa con la Repubblica federale del Brasile. ad esperire, nel prosieguo legale della vicenda, ogni strumento reso disponibile dall'ordinamento giuridico del Brasile per impugnare il diniego all'estradizione, nonché, ove necessario, a ricorrere nelle sedi multilaterali ed europee in tale stessa direzione, anche affinché vengano rispettati i principi di civiltà giuridica che sono alla base dello spazio di giustizia europeo e della stessa Unione europea. Nel quadro delle ottime relazioni tradizionalmente in essere con il Brasile e in parallelo con il percorso giudiziario, si impegna il Governo a mantenere costantemente viva la questione in sede di dialogo politico con il Governo cogliendo l'occasione di tutti i possibili contatti con la nuova Amministrazione per rappresentare alle autorità brasiliane la nostra aspettativa per una corretta interpretazione del contenuto del Trattato bilaterale, e quindi per l'accoglimento dell'estradizione. a farsi interprete dell'auspicio unanime del Parlamento italiano, di fronte al mondo, affinché la soluzione finale della vicenda sia in sintonia con le norme di tale Trattato e con i sentimenti di un'opinione pubblica che, senza distinzioni, è sorpresa e indignata, a volte anche più di chi sta in Senato, per il diniego dell'estradizione, affinché la magistratura faccia quindi la magistratura - ricordiamocelo sempre - e la Corte suprema, mentre pensa ai morti in Italia, confermi ciò che ha sostenuto in 560 pagine di processo.

cari colleghi, intervengo per dichiarare il voto favorevole dell'Italia dei Valori sulla mozione unitaria sull'estradizione in Italia di Cesare Battisti. Come Italia dei Valori abbiamo inteso chiedere che non venisse messa all'ordine del giorno la mozione che come Gruppo abbiamo presentato due anni fa, al fine di poter procedere con un voto trasversale e unitario sul testo frutto del lavoro collettivo dei Gruppi parlamentari, data l'importanza dell'argomento, la necessità di esprimere una posizione forte e unitaria e la volontà di tutti di raggiungere il risultato auspicato. Colleghi, nella lotta al terrorismo non ci sono divisioni, non ci sono ideologismi preconcetti. Allo stesso tempo però, non abbiamo neppure voluto ritirare la mozione dell'Italia dei Valori datata gennaio 2009, perché fosse chiaro all'opinione pubblica, come ai soggetti coinvolti nella dolorosa vicenda, che l'Italia dei Valori sulla questione dell'estradizione di Battisti non è arrivata sull'onda della cronaca di questi giorni, ma da sempre ribadisce con forza la necessità che i cittadini italiani che hanno un gravoso debito con la giustizia e con il loro Paese, come Battisti, tornino nelle patrie galere per scontare ciò che è stato loro comminato dalla magistratura. La giustizia, la legalità, la certezza della pena, il rispetto per le vittime e i loro familiari e la volontà di chiudere un capitolo doloroso della nostra storia,

sul caso Battisti non era così alto, a protestare davanti all'ambasciata brasiliana e, in un incontro ufficioso con l'ambasciatore del Brasile, a chiedere il rispetto della legge e della sovranità dell'Italia. Questa mattina voteremo a favore, in maniera convinta, della mozione unitaria. Lo facciamo per Antonio Santoro, per Pierluigi Torregiani, per Lino Sabbadin e per Andrea Campagna, per il loro ricordo e rispetto, perché la loro memoria faccia in modo che assassinii violenti in nome di una ideologia che professava l'uguaglianza e praticava la morte non avvengano più, per le famiglie che ancora li piangono. Il nostro non è un voto politico, né un voto vendicativo, ma un voto giusto contro chi uccide. Chiederemo altresì che i 113 latitanti italiani che tuttora vivono all'estero, molti dei quali conducono una vita libera e spesso mantengono le fila delle organizzazioni criminali da cui provengono, possano essere riconsegnati alla giustizia italiana, per essere giustamente processati o per scontare le loro colpe nel Paese di appartenenza. Come Italia dei Valori siamo consapevoli che a chiedere il rispetto della sovranità è un Paese democratico, in cui non si viene perseguitati politicamente e la legge è sinonimo di giustizia. Ed è per questa profonda consapevolezza che, quando il ministro della giustizia brasiliano Tarso Genro ha concesso l'asilo politico a Battisti, sulla base di «fondati timori di persecuzione per le sue idee politiche se dovesse essere estradato», ci siamo indignati. indignati. In Italia vige uno Stato di diritto, basato sul rispetto della vita umana, e la nostra concezione della pena, nonostante le difficoltà pratiche nell'applicazione, è fondata non sulle sevizie o sull'umiliazione, ma sulla riabilitazione, percorso questo che non può avviarsi in stato di libertà sulle spiagge di Copacabana. Il Brasile, adducendo queste motivazioni per negare l'estradizione di Battisti, ha di fatto espresso un giudizio negativo sul nostro Paese, sulle nostre forze dell'ordine e sulle nostre istituzioni, un giudizio che non meritiamo e che respingiamo al mittente con questo voto favorevole alla mozione unitaria. Chi tutela i terroristi diventa esso stesso terrorista. il fatto di essere giunti a questo punto, e a dover cercare di porre rimedio alla decisione dell'ex presidente Lula, non può che farci riflettere. In conclusione - ringraziando

ancora ci offende, caro Sottosegretario. Dice infatti Genro che in Italia «questo disagio passerà, come passerà anche il disagio morale di tutti gli italiani davanti al mondo per l'attuale Governo che si ritrovano, e per l'inciviltà e le parole volgari usate da alcuni dei suoi Ministri».

Genro dice: «Voglio solo ricordare al popolo italiano che giustificare l'estradizione di Battisti a partire dalla semplice etichetta di "terrorista", come fanno alcuni esponenti della destra italiana o di altre parti politiche, non serve».

dalla dittatura militare esattamente così, "terroristi", quando in realtà lottavamo per il ritorno alle libertà democratiche».

nostro esame - su una vicenda estremamente grave, non solo per le implicazioni che ha sul piano del diritto internazionale e per la violazione di un Trattato importante, quale quello che regola i rapporti bilaterali tra il nostro Paese ed il Brasile in materia giudiziaria,

delinquente del calibro di Battisti. Si offende poi lo stesso sistema di garanzie costituzionali del nostro Paese e dell'Unione europea, che ovviamente mutua tale sistema. Sono state dette tante cose, che non intendo assolutamente ripetere. Molti colleghi, più autorevolmente e meglio di me, hanno saputo esprimere un sentimento unitario

e i diritti delle vittime dei reati commessi da questo - si fa per dire - signore, siano nelle sedi giudiziarie competenti, brasiliane ed internazionali, tutelati fino in fondo.

all'apertura di un contenzioso giudiziario internazionale, continuare ad intrattenere relazioni bilaterali o commerciali con un Paese che, mentre stringe accordi commerciali con l'Italia, continua a coprire delinquenti e terroristi di questa specie, attribuendo all'ordinamento giuridico italiano una patente di inaffidabilità e contrarietà ai princìpi fondamentali che presiedono alla tutela della persona umana. Signor Sottosegretario, apprezzo molto ciò che lei ha detto e il lavoro svolto dal ministro Frattini, ma dobbiamo essere chiari, e noi intendiamo tornare all'esito delle iniziative, che molto opportunamente, anche su sollecitazione unanime di questo Parlamento, il Governo ha intrapreso e intraprenderà,

amicizia in condizioni di reciprocità, e con l'altra mano, invece, venire ripagati con una patente di inaffidabilità che nega l'estradizione di un delinquente comune. comune. Voglio altresì dire - senza polemica nei confronti del ministro Alfano - che la sottile distinzione (indice di un modo sbagliato di concepire anche la storia e la lettura degli anni di piombo) che distingue il reato politico dal reato comune

che siamo stati vittime, come democristiani, dei peggiori atti di terrorismo in questo Paese, non possiamo legittimare una distinzione tra chi commette un reato per ragioni politiche e chi lo commette per ragioni diverse. Chi commette un reato è un delinquente. Battisti è un delinquente, si è macchiato di una serie di reati,

il percorso giudiziario ma che in maniera quasi pilatesca, ci si lavino le mani affidando al Supremo tribunale e alla Corte internazionale il compito di dirimere questa questione continuando i nostri rapporti garbati

l'errore più grande che il Brasile ha commesso nel negare l'estradizione di Battisti, lo ha commesso anche dal suo punto di vista e dalla sua prospettiva. Questa decisione del presidente Lula rende il Brasile terra di adozione di tutti i peggiori criminali del mondo.

Allora, non solo diventa, dopo Parigi, la seconda patria di quanti hanno commesso delitti, ma altresì la patria di tutti i delinquenti che provengono da Paesi del mondo che nei loro ordinamenti non tutelano questi diritti fondamentali,

decisione demenziale ed irrazionale, che deve farci riflettere su come dobbiamo continuare le relazioni diplomatiche con il Brasile.

Una cosa è certa: il Brasile ci ha dato uno schiaffo micidiale. Ricorderete tutti la sibillina dichiarazione del del 2 dicembre scorso e le affermazioni dell'avvocato difensore di Battisti riguardo alla decisione sull'estradizione, che resero la vicenda ancora più enigmatica. Che cosa voleva dire, come disse lo stesso presidente Lula: «sarà una decisione amara»? sembra riprendere la stessa frase che Mitterrand disse all'emissario del Governo italiano che era andato a perorare la causa dell'estradizione di un terrorista rosso, poi rimasto in Francia Se un Presidente della Repubblica se ne esce con una simile dichiarazione, non viene il sospetto che stava per fregarci? Eppure Lula ha Eppure Lula ha lasciato libero il pluriomicida assassino, oltraggiando i tanti italo-brasiliani e le famiglie delle vittime di Battisti. Si sa, tra ex guerriglieri una certa simpatia può nascere, ed è così che un pluriomicida condannato a tre ergastoli sta per tornare libero, come sembrerebbe in base alle decisione, lo ripetiamo ancora una volta, è uno sfregio alle vittime e alle famiglie distrutte da Cesare Battisti, sicuramente meno interessanti del *business* economico di questo Paese. In questa vicenda, troppe lingue hanno consigliato a Lula di fare rimanere Battisti in Brasile: mi riferisco a un Capo di Stato europeo per il quale era importante non deludere le richieste della consorte, affascinata dai libri del terrorista e menefreghista verso le vittime. Tutti felici, dunque, anche qualche multinazionale a cui conviene che si scambino i morti per inaugurare un nuovo stabilimento e produrre di più. Ho sentito tante preghiere e tanti appelli rivolti a Lula, specialmente da parte della sinistra. Forse bisognava fare come gli israeliani nel 1960, quando andarono in Argentina, impacchettarono Eichmann e se lo portarono a Gerusalemme? È un paradosso, ma non più di tanto. Nessun appello dunque va rivolto al nuovo presidente Rousseff, nessuna preghiera, nessuna supplica e nessuna esortazione. Perché concedere l'estradizione di Cesare Battisti? Semplicemente perché è suo dovere concederla, ed è suo dovere far sì che un terrorista, o meglio un assassino pluriomicida, paghi fino in fondo per le sue colpe di delinquente. Una cosa è certa: per la legge e la giustizia italiana l'oriundo italo-franco-brasiliano Cesare Battisti è inequivocabilmente un assassino, riconosciuto colpevole e condannato a marcire in galera. Il popolo italiano è dalla parte di Abele, e noi non possiamo accettare nessuna decisione che vada contro il popolo e che si basi unicamente su motivazioni ideologiche. Se fosse possibile dirlo con un altro e ben più degno Battisti: ci si emozioni di fronte a un uomo in sedia a rotelle, che ha perso il padre vittima di un agguato e vittima lui stesso. Cari colleghi, è una storia da un certo punto di vista drammatica ma anche paradossale, un miscuglio di mistificazioni, armi e libri gialli, che ha avuto il suo culmine alle ore 18 (ora italiana) del 31 dicembre 2010. Un anno prima, l'operaio metalmeccanico e presidente del Partito dei lavoratori di sinistra, Luiza Inácio Lula da Silva, assicurò a un altro uomo di sinistra, come Giorgio Napolitano, che avrebbe fatto tutto ciò che era possibile per consegnare alla giustizia il sanguinario scrittore di libri gialli e terrorista Cesare Battisti. Non è stato così. È giunto il momento di tirare giù la maschera: siamo stanchi di questi teatrini della politica, ai quali nessuno più crede. Servono azioni e fatti. È necessario restituire alle famiglie delle vittime, e poi agli italiani tutti, la concretezza di tante parole che sono state spese e profuse per celare comportamenti che lasciano trasparire quanta meschinità, incapacità e pochezza esiste in tutti coloro che, a vario titolo, hanno gestito la vicenda Battisti. Non vorremmo lasciare ai nostri figli l'immagine del nostro Paese servo del Brasile.

da decenni Cesare Battisti, dopo aver commesso in Italia gravissimi delitti comuni, si sottrae alla giustizia italiana. Gli ultimi tre anni di latitanza li ha passati in Brasile. Dico subito che considero grave la decisione del Brasile di non concedere l'estradizione per Battisti. Grave perché viola illegittimamente il trattato di estradizione tra Italia e Brasile, viola la decisione del supremo Tribunale brasiliano e perché viola i principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. È grave anche perché Battisti è stato un criminale comune, sino al momento in cui considerò più utile trasformarsi in un delinquente politico e atteggiarsi a perseguitato per motivi politici. È su questa mistificazione che Battisti ha costruito la sua difesa, sempre lucrandone ogni possibile tornaconto. Un segnale che la misura è colma viene persino dalla recentissima decisione, proprio del Brasile, di revocargli la qualifica di rifugiato politico. Dico tutto ciò subito perché questo è il senso politico della mozione che i senatori del Partito Democratico tra breve voteranno, ed è anche il mio personale pensiero. Considero un atto di responsabilità e di serietà del Senato che la mozione sia stata sottoscritta dai Gruppi della maggioranza e dell'opposizione, a conferma che vi sono questioni sulle quali non è corretto assumere posizioni politiche di pura contrapposizione partigiana. L'Italia è tradizionalmente amica del Basile e i senatori del Partito Democratico vogliono che il buon rapporto tra i due Paesi prosegua e si consolidi. È proprio questa solida amicizia che ci obbliga ad esprimere, con lealtà, un giudizio severo e franco sulla mancata concessione dell'estradizione. Ma la vicenda Battisti, signor Sottosegretario, non parla solo di un consistente errore politico di un grande Paese come il Brasile. Parla molto anche di noi, della storia dei nostri anni '70 e '80, di cui ha parlato molto bene poco fa il senatore Tonini, e anche della nostra storia attuale. Ha ragione il Presidente della Repubblica quando ricorda che il nostro Paese non è riuscito a far capire, anche a Paesi amici, cosa abbia significato per noi il terrorismo degli anni '70 e '80 e quanto sia stato importante per la nostra democrazia riuscire a sconfiggerlo senza leggi speciali e tribunali speciali. Sono stati per l'Italia anni molto difficili, ma anche anni nei quali i princìpi fondanti della Repubblica erano custoditi da partiti grandi e piccoli che, pur tra tanti errori, hanno saputo resistere alle tentazioni populiste e alle derive giustizialiste. Anni che hanno visto grandi *leader* vivere con decoro, onore, dignità e senso del limite. Alcuni di loro sono stati colpiti anche da pesanti inchieste giudiziarie, ma mai nessuno ha detto che i giudici sono una metastasi della democrazia. Negli anni '70 l'Italia non ha violato né i valori della separazione dei poteri né quelli dello Stato di diritto, e non lo ha fatto nemmeno per battere il terrorismo, mentre oggi li si viola per bassi interessi politici. Tutto questo travaglio l'Italia non è riuscita a suo tempo a spiegarlo nemmeno alla Francia di François Mitterrand. Non ci sono riusciti i Governi e non ci sono riuscite le forze politiche di centro, di sinistra e di destra. Ma chi ha personalmente assistito ai tre incontri che negli ultimi anni il presidente Berlusconi ha avuto con il presidente Lula sa che che in quelle occasioni mai l'onorevole Berlusconi ha richiesto esplicitamente con forza l'estradizione di Battisti, mai ha sostenuto personalmente con chiarezza la necessità che il Brasile onorasse i trattati con l'Italia e mai ha chiesto al presidente Lula un esplicito impegno politico. omissioni italiane nulla tolgono all'errore della mancata estradizione, ma è possibile che questo silenzio sia stato valutato e che le richieste della nostra diplomazia non siano state adeguatamente considerate. La mancata estradizione di Battisti accresce il dolore dei parenti delle vittime del terrorismo e offende tutti gli organi dello Stato, che per tanti anni hanno lottato contro il terrorismo con le armi del diritto e della democrazia, ma la dice anche lunga su quanto sia profonda la perdita di prestigio e autorevolezza internazionale del nostro Governo e quanto gravi possano esserne le conseguenze. *(Applausi una nuova finestra"). È presente in Aula una delegazione dell'Istituto comprensivo «Sandro Penna» di Battipaglia, in provincia di Salerno. A loro va il saluto dell'Aula.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, Cesare Battisti è un delinquente comune, un volgare assassino, che disonora un nome a noi particolarmente caro che ci riporta all'indimenticabile martire risorgimentale. Battisti fu per la prima volta arrestato nel 1972, per una rapina compiuta a Frascati. Nel 1974 venne nuovamente tratto in arresto per una rapina con sequestro di persona, quella volta compiuta a Sabaudia. Dopo aver raggiunto la maggiore età, nel 1977 fu arrestato, sempre per rapina, e rinchiuso nel carcere di Udine dove entrò in contatto con Arrigo Cavallina, ideologo dei Proletari armati per il comunismo, che lo accolse nell'organizzazione. Trasferitosi a Milano, iniziò a partecipare alle azioni del gruppo eversivo, responsabile prima di varie rapine a banche e supermercati nel quadro di quelli che venivano definiti espropri proletari e successivamente anche di alcuni omicidi di commercianti e appartenenti alle forze dell'ordine. In Italia Cesare Battisti è stato condannato come responsabile di quattro omicidi. Queste sono le date, scolpite nella nostra memoria e che nessuno di noi deve dimenticare per doveroso rispetto alle vittime ed affettuosa, convinta solidarietà alle loro famiglie: 6 giugno 1978 a Udine, Antonio Santoro, maresciallo della Polizia penitenziaria; 16 febbraio 1979 a Milano, Pierluigi Torregiani, gioielliere; 16 febbraio 1979 a Santa Maria di Sala, Lino Sabbadin, macellaio; 19 aprile 1979 a Milano, Andrea Campagna, agente della Digos. Nel 1979 Battisti fu arrestato e tradotto nel carcere di Frosinone, da dove il 4 ottobre 1981 riuscì ad evadere e a fuggire, prima in Francia, quindi in Messico, poi nuovamente in Francia. Il Consiglio di Stato francese e la Corte di cassazione transalpina, con due successive decisioni sulla richiesta di estradizione, autorizzarono la consegna di Battisti alle autorità italiane. Battisti si rese però latitante, lasciando la Francia e facendo perdere le sue tracce. Un ultimo ricorso, presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, contro la sua estradizione in Italia, venne dichiarato dalla stessa Corte inammissibile nel dicembre del 2006. Fu quindi arrestato a Copacabana, in Brasile il 18 marzo 2007, a seguito di brillanti indagini congiunte di agenti francesi e carabinieri del ROS. Il 13 gennaio 2009 il Brasile ha deciso di accordare lo *status* di rifugiato politico a Cesare Battisti. Il ministro della giustizia Tarso Genro ha motivato tale davvero inaccettabile decisione su quello che definisce il fondato timore di persecuzione del Battisti per le sue idee politiche, nonché sui dubbi espressi sulla regolarità del procedimento giudiziario nei suoi confronti. La decisione del Governo brasiliano ha giustamente suscitato aspre reazioni sia da parte del Governo italiano e del suo presidente Berlusconi, sia da parte dell'opposizione di centrosinistra, sfociate nella mozione *bipartisan*, approvata all'unanimità dal Parlamento, per richiedere la revoca dello *status* di rifugiato politico dell'ex terrorista. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha in seguito inviato una lettera al suo omologo Luiz Inácio da Silva in cui ha espresso il proprio stupore e rammarico per la decisione del Governo brasiliano: stupore e rammarico che sono dell'intero popolo italiano. Sulla decisione brasiliana è da ultimo intervenuto il Parlamento europeo, che ha approvato una risoluzione che chiede al Governo dello Stato sudamericano di tenere conto delle sentenze italiane sul caso Battisti. Il 31 dicembre dell'anno scorso l'ex presidente Lula annuncia il proprio rifiuto all'estradizione di Battisti in Italia, seguendo l'inaccettabile orientamento dell'Avvocatura di Stato brasiliana. Il Supremo Tribunal Federal, la Corte costituzionale brasiliana, conferma però la legittimità della carcerazione di Battisti sino alla sua definitiva pronuncia. Questi sono i fatti, davvero incontestabili. È quindi davvero indispensabile che il Governo italiano percorra tutte le strade possibili, nessuna esclusa, perché venga rimosso dalla Corte suprema brasiliana l'incomprensibile ed ingiusto rifiuto dell'ex presidente Lula alla concessione dell'estradizione e Cesare Battisti possa finalmente scontare in Italia le pene detentive a lui irrevocabilmente inflitte per tutta una serie di efferati crimini comuni. altresì necessario qualsiasi ulteriore intervento volto ad impugnare il diniego all'estradizione, ricorrendo a tutte le sedi europee ed internazionali, per assicurare il rispetto dei princìpi di civiltà giuridica che sono, o dovrebbero essere, alla base dei valori universali dell'intera umanità. È importante denunciare all'opinione pubblica europea, così come detto nella mozione al nostro esame, che il provvedimento del Governo brasiliano mette in discussione il rispetto dei princìpi stessi di civiltà giuridica da parte di tutta l'Unione europea, quale omogenea comunità di valori e spazio di libertà e giustizia, essendone l'Italia un Paese membro. Bisogna Bisogna altresì in tutte le occasioni di incontri istituzionali rappresentare alle autorità brasiliane la nostra ferma aspettativa per l'accoglimento di una estradizione fortemente voluta dall'intera opinione pubblica italiana, senza distinzioni di parte, particolarmente indignata per gli ultimi sviluppi di una vicenda che vede coinvolto un assassino, un delinquente comune, come tale riconosciuto da sette processi e da 24 giudici italiani. Il Gruppo del Popolo della Libertà voterà quindi convintamente a favore della unanime mozione illustrata dal senatore Compagna, a testimonianza di un impegno comune per indurre un Paese, che si dice amico e che noi vogliamo tale, quale la Repubblica Federativa del Brasile, ad uniformarsi alle sacrosante ragioni dello Stato e del popolo italiano.

contratto è molto importante in quanto prevede una rappresentazione dell'immagine femminile molto più rispettosa della sua dignità e un codice deontologico proprio su questo